Il seguito della settimana corrente sarà riservato ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento ai decreti-legge presentati al Senato. La prossima settimana, martedì 10, alle ore 16,30, e nella giornata di mercoledì 11 novembre sarà discusso il decreto-legge recante proroga misure di contrasto al Covid-19. Giovedì 12 novembre, alle ore 9,30, è previsto il *question time* con la partecipazione dei Ministri per gli affari europei, dello sviluppo economico

Onorevoli senatrici e senatori, nella giornata di ieri una serie di attacchi terroristici ha colpito la città di Vienna, causando vittime e feriti tra cittadini inermi e Forze di polizia. L'aggressione violenta, vile, in disprezzo della vita delle persone, della storia e della cultura di una delle capitali dell'Europa, rappresenta, non solo una ferita profonda per Vienna, per l'Austria e per il suo popolo, ma anche una inaccettabile minaccia verso i valori e i diritti fondamentali della civiltà e della democrazia. Nessuna ragione, nessuna ideologia, nessuna attenuante possono giustificare condotte che rappresentano crimini contro la stessa umanità. Di fronte al dolore, allo smarrimento, alla privazione violenta della libertà deve levarsi, unanime, la risposta comune, fondata sulla condanna senza incertezze di ogni intimidazione e violenza e, allo stesso tempo, sulla piena solidarietà e vicinanza alle vittime innocenti e all'Austria intera, verso la quale oggi ci sentiamo ancora di più stretti da legami e sentimenti di autentica amicizia. In ricordo delle vittime, con gratitudine verso i soccorritori e in spirito di partecipazione verso i cittadini e le istituzioni austriache, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, come Gruppo per le Autonomie e rappresentanti della SVP, esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle istituzioni e al popolo austriaco per i fatti di ieri sera. Ci sentiamo particolarmente vicini alle famiglie delle vittime. Sono antichi e profondi i legami del Sudtirolo con la città di Vienna; un'amicizia che, mai come oggi, avvertiamo la necessità di sottolineare e di ribadire. Quanto è successo avviene a pochi giorni dagli attentati in Francia. Fa riflettere la strategia del fondamentalismo islamista di creare scompiglio e terrore in una fase in cui l'Europa tutta è chiamata a fronteggiare la drammatica emergenza sanitaria. È l'ennesima riprova, semmai ce ne fosse stato bisogno, di un disegno malato e disgustoso, cui l'Europa deve rispondere in maniera unitaria, rilanciando il suo impegno contro ogni forma di fondamentalismo e di intolleranza. Il terrorismo ci fa paura, sì, ma, nello stesso tempo, aumenta la nostra fermezza per la scia di dolore e morte che semina tra tanti cittadini inermi e innocenti, la cui unica colpa è di di essersi trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Questo, per tutti noi, è semplicemente inaccettabile. Chi semina il terrore, chi vuole trasformare le nostre città in scenari di guerra deve, però, sapere che l'Europa, nella sua storia, ha saputo sconfiggere avversari molto più grandi e più minacciosi. Quindi, lo farà anche questa volta, per onorare le vittime di una guerra che esiste soltanto nelle menti disturbate di chi calpesta e manipola un messaggio religioso per perseguire scopi che nulla hanno a che fare con la fede e con la religione. Viva la libertà! Viva il popolo austriaco, cui, da quest'Aula, mandiamo l'abbraccio più grande e più commosso di cui siamo capaci.

alle istituzioni austriache, ai familiari delle vittime, alle Forze dell'ordine e a tutta la cittadinanza austriaca. Un nuovo attacco, che non è un attacco solo all'Austria, ma all'Europa tutta, tra l'altro a pochi giorni dagli altri avvenimenti che avevano riguardato prima Samuel Paty, l'insegnante francese sgozzato brutalmente, e poi successivamente Nizza, ancora teatro di sanguinosi omicidi. omicidi non arrivano dall'Islam - è importante ribadirlo fortemente proprio all'interno delle istituzioni - ma da terroristi islamici, terroristi islamici, che ci devono vedere uniti a livello europeo e convintamente volti a contrastare queste forme di brutale e fanatica violenza.

un'agenzia estremamente proficua che ha dimostrato anche nei recenti attentati, che purtroppo hanno a loro volta insanguinato le principali capitali europee, di essere uno strumento importante e prezioso. È necessario che a livello europeo adesso si potenzino strumenti come questo, cosa che invece non è stata fatta nella recente proposta della Commissione europea rispetto al bilancio.

modo, è necessario potenziare lo scambio delle banche dati, prevedere una formazione a livello internazionale per le forze inquirenti sia di magistratura che di polizia che di polizia e rafforzare le squadre investigative comuni. Anche a livello nazionale è necessario che ci si doti di leggi e si recepiscano le diverse decisioni e direttive europee finalizzate a migliorare la collaborazione a livello internazionale e, in particolare, comunitario

e quanto siamo per una concezione liberale dello Stato. Nell'esprimere la nostra profonda solidarietà, questa deve essere anche un'occasione per ribadire un impegno politico forte, oltre che di potenziamento degli strumenti idonei al contrasto del terrorismo. (*Applausi*).

all'Austria, ai cittadini e alle vittime di questo ennesimo attentato terroristico tutta la sua solidarietà di italiani ed europei. È purtroppo triste constatare che in pochi giorni in quest'Aula abbiamo dovuto esprimere la nostra solidarietà alle vittime e al popolo francese per due volte e ora al popolo austriaco.

Noi gliene diamo atto perché pensiamo che sia assolutamente necessario, oggi più che mai, ritrovarci insieme nella consapevolezza di quale sia il fenomeno terroristico che colpisce nel cuore

È uno scontro di civiltà, anzi è l'assalto alla civiltà di chi non ha civiltà. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo: è l'assalto alla civiltà cristiana, giudaica e latina; è l'assalto alla civiltà laica che ha fondato sulle libertà la crescita e lo sviluppo del nostro continente, insegnando agli altri la strada su cui incamminarsi. Dall'altra parte, nel fondamentalismo islamico, non certo nell'Islam, non c'è una civiltà, c'è l'odio nei confronti delle civiltà e, quindi, anzitutto l'odio nei confronti della nostra civiltà.

e solo noi forse riusciamo a sancire), le scuole e la libertà di insegnamento, lo spirito critico, satirico e dissacrante, che è poi creativo e a fondamento dell'arte, della cultura, del sapere, della crescita dell'umanità e di ciascuna persona che ne fa parte. Loro sono i nemici di tutto questo e noi dobbiamo difendere tutto questo perché è fondamento del nostro agire comune. Hanno colpito anche, certo, i luoghi della gioia, dello svago, della mondanità. Anche la gioia, lo svago e la mondanità, insieme alla religione, alla scuola e alla formazione, fanno parte della civiltà della luce e della dignità che è la nostra civiltà, mentre la loro appartiene alla violenza delle tenebre e dell'oscurità. Proprio perché sappiamo che c'è questa contrapposizione in atto, noi dobbiamo essere uniti, come italiani e come europei, ma dobbiamo anche reagire non soltanto accomunandoci nella solidarietà e nella commemorazione. Dobbiamo reagire ben consapevoli che l'Italia è la frontiera di tutto questo. È la frontiera, come dimostra il caso ripetuto di Lampedusa, ma è anche il cuore della civiltà europea. Per tali ragioni vi chiediamo di agire per chiudere quella frontiera, per chiudere il porto di Lampedusa se è il simbolo della rotta del terrore. Vi chiediamo insieme di reagire, perché soltanto reagendo insieme nelle misure comuni, noi sapremo dimostrare loro, che ci colpiscono nel cuore e nel cervello, che siamo la civiltà e, come tale, andremo avanti e vinceremo la sfida delle tenebre.

Signor Presidente, anche noi ovviamente ci uniamo al dolore e al cordoglio per le vittime di questo attacco terroristico e lo facciamo come Gruppo Misto, come componente di Liberi e Uguali. Credo sia, come si sta dimostrando in questa discussione, un sentimento condiviso tra colleghi e tra i nostri connazionali. È stato un attacco vile, vigliacco, perché non solo avviene a pochi giorni dai fatti di Nizza, da quella vicenda orribile e inquietante che ha toccato la città di Parigi, che è stata ricordata, ma perché accade e cade a poche ore dalla serrata a cui si accingeva la città di Vienna. Avviene quindi nel cuore di un'Europa già sotto assedio, spaventata e impaurita in ragione di una guerra contro un altro nemico, altrettanto subdolo e invisibile: il virus, che sta mettendo a dura prova non solo i corpi delle donne e degli uomini di questo continente, ma soprattutto la tenuta persino psicologica dei nostri concittadini e dei cittadini di questo continente e di tutto il mondo. Da questo punto di vista è un attacco deprecabile che noi dobbiamo condannare senza se e senza ma, senza giustificazionismi sociologici o di altra natura. Stiamo parlando di persone difficilmente annoverabili nel genere umano che hanno attaccato e ucciso innocenti.

ad uscire dalla rappresentazione che ha dato il cancelliere federale austriaco Sebastian Kurz - che non è propriamente in sintonia con la mia sensibilità politica, anzi, è quanto di più distante dalla mia idea di politica - il quale ha detto, poche ore fa, che non siamo di fronte alla contrapposizione tra il mondo cristiano e il mondo musulmano, non stiamo parlando di questo e non dobbiamo parlare di questo, perché se noi diamo l'idea che questa è la rappresentazione che diventa l'oggetto della nostra discussione, facciamo esattamente il gioco di quei terroristi che vogliono che quella rappresentazione sia la dimensione reale, la fotografia della realtà. *(Applausi)*. È in ragione di tale rappresentazione che agiscono sulle leve che noi dobbiamo neutralizzare, che dobbiamo eliminare e che stanno dentro la società europea, nel cuore della società europea. Infatti, Presidente, ci sono due cose che noi non possiamo dimenticare: l'Europa non è una fortezza che deve erigere dei muri e dentro la quale cresce automaticamente un'idea di democrazia. Come tutte le grandi democrazie, l'Europa vive nelle e delle sue contraddizioni e se noi non andiamo a vedere innanzitutto dove si annidano quelle contraddizioni, fatte anche di condizioni materiali e di disuguaglianze, che sono esattamente le leve

che dobbiamo tenere in considerazione: l'Europa deve ritrovare il senso di un rapporto con il resto del mondo. Noi non possiamo essere permanentemente in guerra con il mondo, dalla Russia all'Iran, passando per la Turchia, facendo finta di non saper distinguere neanche più che all'interno dello stesso mondo islamico esistono il mondo sciita e il mondo sunnita con un'articolazione molto complessa. Quindi, recuperare il senso della politica, il senso di una strategia nelle relazioni internazionali, vuol dire anche capire

vile attentato di queste ore, come quelle che abbiamo commemorato - ahimè - soltanto pochi giorni fa. Signor Presidente, Vienna dopo Nizza, due città europee che sono nel pieno della storia del nostro continente, aperte al mondo e forse per questo prese di mira, come il nostro modello di vita e il nostro insieme di valori, città ancora insanguinate. L'orrore ci ha colto all'improvviso anche l'altra sera, come è stato per Nizza, quindi voglio aggiungermi alla solidarietà e alla vicinanza espressa da lei, Presidente, per portare l'abbraccio del Gruppo Partito Democratico alle famiglie delle vittime, a tutto il popolo austriaco a tutto il popolo austriaco e, se mi permette, in particolare alla comunità ebraica, che è stata probabilmente presa di mira, e anche alla comunità araba islamica, quella onesta, che ha deciso di fare di quel posto la sede della propria vita, paga il prezzo di questi eventi che rischiano di mettere in difficoltà e di interrompere i percorsi di integrazione. *(Applausi)*. Nella storia europea la dignità della vita umana è al primo posto e nella nostra Carta, nella stessa Carta europea, sono scolpiti i valori della libertà di espressione, di opinione politica, di religione, di espressione dei propri orientamenti sessuali. Questa è la nostra storia e non dobbiamo non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo: non possiamo rinnegare la nostra storia. Quindi nel nostro continente non accetteremo mai che usino l'odio religioso come scusa per le loro azioni deplorevoli. Su questo faremo sempre fronte comune: non possono utilizzare la religione per giustificare le loro azioni atroci. Chi commette questi atti - e lo diciamo ai più giovani, anche delle comunità islamiche - non è un martire, è un criminale e questo deve essere chiaro a tutti i livelli.

guida di un Governo di destra, ha detto in maniera molto chiara che non è una guerra tra cristiani e islamici, non è una guerra fra austriaci e migranti, ma è una guerra tra fra chi vuole la pace e i pochi

Farci chiudere, tuttavia, rinunciare alla nostra storia e alle nostre libertà è proprio l'obiettivo di quei terroristi e a questo atteggiamento ci dobbiamo evidentemente ribellare. Non basta solo questo, è evidente, perché servono interventi sociali, culturali, oltre ad interventi dal punto di vista della sicurezza e non bastano le mere misure nazionali. Oggi noi vinciamo, se abbiamo una risposta a livello europeo, a livello culturale e di solidarietà. Quando siamo colpiti, non è che siamo tutti francesi o tutti austriaci: siamo tutti europei e servono misure a livello europeo. Riprendo uno dei punti sollevati dalla senatrice Garavini: noi abbiamo una sfida molto importante. Abbiamo fatto grande fatica per affermare la procura europea

delle infiltrazioni della criminalità organizzata e del terrorismo di matrice islamica. Ebbene, penso sia giunto il momento di fare un salto di qualità, di non avere timori e indugi. Credo che questa sia una battaglia da fare tutti insieme, che tutti i senatori tutti i deputati possano sostenere lanciando un messaggio molto chiaro: abbiamo bisogno di misure europee per affrontare il terrorismo internazionale. No, quindi, alle scorciatoie sovraniste e sì, invece, ad un'Europa più forte per sconfiggere e affrontare quelle sfide che oggi non siamo più in grado di sostenere da soli.

abbiamo ascoltato parole forti di sdegno da parte della Presidente della Commissione europea, del commissario Gentiloni Silveri e di altri, ma sono parole

Non sono ancora chiari tutti i fatti: leggevo poco fa che in Austria un Ministro ha contestato il comportamento del protagonista dell'attentato di Vienna, che avrebbe ingannato - non so ancora in quali modi - i programmi di deradicalizzazione

a me ha colpito molto in questi anni che quasi sempre - per ora non l'abbiamo ancora ben capito per Vienna - per tutti i protagonisti degli attentati, se ci avete fatto caso, dopo pochi minuti o poche ore si conosceva la loro storia,

hanno costellato il mondo di tragedie erano stati schedati e individuati come fondamentalisti. Allora è tempo o no di un'azione preventiva, anche di fermo, di coloro che, conosciuti, non possono essere lasciati liberi fino a quando non decidono di uccidere, dietro l'angolo, il primo che passa? È una scelta dura, ma che forse va ipotizzata, perché molti di questi personaggi poi finiscono uccisi

Se li si trattenesse prima, forse la pena per loro sarebbe più lieve di quella a cui poi vanno incontro. L'Europa si deve dunque porre questo problema: se si conoscono persone fomentano l'odio e che si sono oramai inserite in un'attività non di diritto religioso, ma di radicalismo religioso, che prepara stragi, forse servono norme come quelle che l'Italia democratica ha emanato negli anni del terrorismo del terrorismo interno. Abbiamo affrontato quegli anni con leggi speciali, che in tempi ordinari non si farebbero. Vedo che anche in Francia, l'altro giorno, il Ministro di un Paese che fa della democrazia e della libertà il proprio vanto, parlava di una Guantanamo europea. Dobbiamo anche chiarire a livello internazionale, cari colleghi, la posizione della Turchia, un Paese che abbiamo considerato amico e che fa parte della NATO. La Turchia ci deve spiegare se fiancheggia e spalleggia tentazioni fondamentaliste, dalla Libia ad altri luoghi del Nord Africa e dell'Oriente, o se vuol far parte addirittura dell'Unione europea, oltre che della NATO: ci sono ambiguità. Vienna è, peraltro, un luogo simbolico: assediata alla fine del Seicento, fu teatro di uno degli scontri epici di civiltà. Possiamo negarlo o meno, ma c'è anche uno scontro

Oggi l'Egitto è un baluardo contro il terrorismo. Qualcuno in Italia invece lo considera quasi un Paese nemico da boicottare. Cominciamo dunque a dire queste cose a stare anche attenti in Italia. Non tutti quelli che sbarcano sono terroristi, lo sappiamo bene, ma sbarcano anche dei terroristi. In Italia si processa chi blocca gli sbarchi e si dà accoglienza e protezione a chi, sbarcando, prepara omicidi in giro per l'Europa.

blocchi gli ingressi di clandestini *(Applausi)*. Altro che smantellamento dei decreti! Basta retorica, colleghi! Siamo assediati e l'assedio impone una risposta di civiltà, ma anche di fermezza.

perché, signor Presidente, è certamente vero che non tutti gli islamici sono terroristi, ma non si può ignorare che questi terroristi sono tutti islamici. Non si può ignorare, signor Presidente, al netto del non volere fomentare lo scontro di civiltà, che oggi c'è una Turchia tutt'altro che laica, che fomenta lo scontro di civiltà. Non si può ignorarlo, anche nella gestione dei rapporti tra l'Europa e la Turchia, perché se in Francia le cose sono accadute, una responsabilità va cercata ad Ankara. Le responsabilità vanno prese e dobbiamo essere forti. Lo dico al senatore La Forgia che è intervenuto prima di me dicendo che l'Europa non ha mura, non ha una fortezza da difendere. Sì che ce l'ha ed è fatta di valori, di identità, di cultura, di secoli di libertà professata. Qualcuno ha armato la mano di questi che sono pazzi, perché ovviamente sono sempre pazzi (se va ad ammazzare, una persona non può essere sana di mente); quando ammazzano nel nome di Dio, nel nome di Allah, lo fanno perché qualcuno ha armato la loro mano. Non so se riusciremo mai a disarmare quella mano, ma so che noi abbiamo dei valori da proteggere e so che se queste mura fatte di valori non vengono mantenute si sgretolano. Allora non possiamo rinunciare a questi valori; in nome di una melassosa accoglienza indiscriminata, non possiamo negare che ci sia una differenza culturale di base,

Signor Presidente, ci sono anche delle cose che ci sconcertano e sulle quali abbiamo bisogno di rassicurazione, come il fatto di scoprire che quel terrorista di Nizza era dei tanti cosiddetti i profughi sbarcati a Lampedusa che profughi non sono, ma che come abbiamo potuto vedere poi si armano e uccidono le persone. In questi tre giorni sono sbarcate più di 2.000 persone a Lampedusa,

C'è fatica a dire che chi sta sbarcando a Lampedusa è a rischio di infiltrazioni in Europa per l'Islam; c'è fatica a riconoscere queste cose *(Applausi)*. Noi abbiamo bisogno e chiediamo al Governo di avere sicurezza. Chiediamo di difendere questi valori, signor Presidente, perché altrimenti anche quel sangue sarà stato versato per niente e saremo qui ancora domani a fare commemorazioni e questo non lo vogliamo. Abbiamo delle mura forti e benfatte d'identità, di cultura, di storia e di libertà, le vogliamo difendere? Quello che Quello che voi ci proponete è il sonno della ragione. Noi invece diciamo: sveglia, il tempo sta scadendo! Sveglia, difendiamo queste mura di libertà! Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle si stringe ai viennesi in queste ore drammatiche esprimendo loro la massima solidarietà e vicinanza, in particolare ai familiari delle vittime di questo nuovo orrendo attacco che torna a colpire l'Europa. Quest'Assemblea è con voi e non vi lascia soli. La violenza terroristica che usa la religione come pretesto per seminare paura nella nostra società, già sfibrata dalla crisi causata dalla pandemia, rischia di destabilizzare le nostre democrazie soffiando sul fuoco dell'intolleranza e dell'estremismo politico. Per questo rappresenta un nemico che va combattuto con freddezza e lucidità, senza alimentare ulteriormente paura e odio, senza strumentalizzazioni. Come ha dichiarato oggi il ministro degli affari esteri Di Maio, è obiettivamente necessario e urgente migliorare i controlli su chi entra in Europa e, quindi, la condivisione di *intelligence* con i Paesi d'origine per evitare l'ingresso e la permanenza sul nostro territorio di lupi travestiti da agnelli, di terroristi che si mischiano ai migranti e ai rifugiati con lo scopo preordinato di compiere attentati, come accaduto per il tunisino Quanto accaduto a Vienna, invece, almeno dalle informazioni finora disponibili, ha a che fare con il problema della radicalizzazione degli immigrati di seconda generazione. L'attentatore di Vienna è, infatti, un cittadino austriaco ventenne nato in Austria da una famiglia di origine albanese macedone, che si è radicalizzato fino ad affiliarsi all'Isis. Ecco quindi la necessità di investimenti in integrazione, ma anche di maggiori controlli su moschee, centri culturali, associazioni nelle quali si fa propaganda e proselitismo fondamentalista. Questo vuol dire una migliore *intelligence* su certi ambienti, come quelli collegati al movimento internazionale della Fratellanza musulmana, realizzata con l'indispensabile collaborazione delle nostre comunità islamiche moderate e dei Paesi islamici, da cui partono finanziamenti a queste organizzazioni. In conclusione, consentitemi una riflessione di prospettiva, nella speranza che quanto sta accadendo ci serva per non ripetere in futuro gli errori del passato. Sappiamo tutti, infatti, come l'Occidente, che oggi è sotto attacco da parte di questi criminali, abbia soffiato per decenni sul fuoco dell'integralismo islamico, quando questo era utile ai nostri scopi geopolitici in Afghanistan, nel Caucaso, nei Balcani, in Medio Oriente e in Nord Africa. Presidente, è nostra responsabilità storica richiudere nella lampada il genio malefico che purtroppo abbiamo contribuito a liberare e che ora minaccia tutti noi.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

Signor Presidente, desidero intervenire al termine della seduta, sperando di avere l'attenzione di tutti i colleghi, per un fatto molto grave. In queste ore, che dovrebbero vedere impegnato il Governo a fronteggiare la seconda ondata di emergenza sanitaria, dovuta all'inconsistenza di ciò che è stato fatto in questi mesi, fonti di stampa hanno anticipato una bozza di decreto-legge che riguarderebbe la scellerata decisione di prolungare il commissariamento della sanità in Calabria. Al di là del fatto che un nuovo decreto Calabria (ricordo ancora il primo: una scatola cinese di un commissario, con un subcommissario, con un vice subcommissario) è uno spreco enorme di soldi, sottratti alla sanità calabrese,

affermato che esso costituiva un intervento normativo non ordinario, ma straordinario, per affrontare con determinazione e rapidità il tentativo di traghettare la sanità calabrese verso situazioni di normalità. Presupposto comunque che l'evidenza non è questa, in questo momento la Regione Calabria, a seguito delle elezioni del gennaio 2020, ha intrapreso un percorso virtuoso, volto a ricondurre la gestione del servizio sanitario regionale a canoni di efficacia ed efficienza. A maggior ragione, commissariarla adesso, quando è stata praticamente individuata come zona rossa, significa toglierle i mezzi per combattere una guerra. L'emanazione di un nuovo decreto-legge di commissariamento finirebbe per ledere gravemente le competenze regionali in materia di tutela della salute. Noi tutti non possiamo e non dobbiamo dimenticare che i commissari governativi che si sono alternati negli ultimi dieci anni avrebbero dovuto ricostruire, ancor prima che risanare, il governo della salute in Calabria. Invece, tutti questi commissariamenti hanno soltanto aumentato la spesa regionale. E si vuole prolungare e rinnovare il provvedimento? Bravi. La gestione commissariale della sanità calabrese va avanti da dieci anni. Dieci anni in cui è peggiorata la qualità dei servizi erogati e sono aumentati i viaggi della speranza.

A me stupisce che uno dei partiti di maggioranza, espressione politica proprio dei presidenti Zingaretti e De Luca, quasi neghi un modello vincente per puntare su un modello commissariale che ha fallito per dieci anni.

per l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria da finanziare ex articolo 20 e degli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute: una partita che supera il miliardo di euro di fondi in parte impegnati, in parte da impegnare, ma sicuramente da spendere.

in cui la pandemia sta cambiando e sconvolgendo le nostre relazioni e il nostro vivere sociale, vorrei portare alla vostra attenzione una storia che nella sua semplicità e ordinarietà, ma con la sua profonda umanità, deve farci riflettere e dare lo spunto per alcune semplici considerazioni. Di situazione analoghe sicuramente nel nostro Paese ne avvengono quotidianamente, anche se con motivazioni diverse tra loro, ma tutte sono accomunate da un unico comune denominatore: il grande cuore di tanti nostri concittadini. Un medico pediatra di Napoli, il dottor Eduardo, viene chiamato a visitare presso la propria abitazione una piccola bambina ammalata; la sua famiglia vive con profonda dignità ed animo semplice le sue gravi difficoltà economiche, acuite dall'emergenza del momento. Ebbene, il dottor Eduardo, ben comprendendo le oggettive ed evidenti problematiche familiari, presta la sua opera con professionalità, ma rifiuta qualsiasi riconoscimento economico: azione questa che, nel rispetto del giuramento d'Ippocrate, rappresenta la dimostrazione di come molto spesso, anche nei semplici gesti, l'animo umano riesce ad esprimere il meglio di sé. Il dottor Eduardo fa semplicemente quello che ogni medico fa normalmente e quotidianamente: rispondere alla domanda di salute di ogni cittadino, immedesimandosi però al tempo stesso nelle sue problematiche sociali. Ciò rappresenta il compito gravoso che tantissimi operatori sanitari, in modo diverso e qualificante, svolgono con competenza, professionalità ed umanità, in molteplici e difficili contesti ambientali. Si può essere i migliori professionisti per competenze, ma senza umanità o empatia con il paziente non si potrà mai aiutare *in toto* chi è ammalato e necessita del nostro aiuto professionale. Il paziente viene prima di tutto e di tutti. I medici non devono essere considerati eroi, ma semplicemente uomini nell'animo e nelle azioni. Concludo, Presidente: la particolare attenzione data alle persone più fragili o più deboli non deve rappresentare l'eccezione, ma la regola e la normalità, sia nella professione medica, sia in generale nella vita di una collettività. *(Applausi)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, è un momento di grande difficoltà per il nostro Paese - inutile ribadirlo anche una fase molto importante e abbiamo l'enorme responsabilità di gettare le basi per una ripartenza e per il futuro dell'Italia. Nella drammatica crisi che stiamo vivendo ci sono sfide e opportunità che abbiamo il dovere di raccogliere, perché alcuni processi di cambiamenti epocali stanno accelerando il loro percorso in una società sconvolta, che vede maturare i propri paradigmi. Uno dei modelli che sta velocemente cambiando è quello del settore energetico: tutti i più grandi Paesi stanno completando la loro transizione energetica dalle fonti fossili verso le fonti rinnovabili.

delle aree idonee, lo testimoniano. La mancanza di questo piano energetico nazionale è un problema che si ripercuote negativamente su diversi livelli: genera incertezza e blocca le iniziative dei privati; crea conflitti e divisioni sui territori e gli enti locali vanno in ordine sparso con approcci disomogenei. Il Governo deve avere un ruolo determinante; non possiamo perdere tempo. È un allarme che lancio a questo Governo, che sostengo; ci sono tanti altri aspetti sui quali sta agendo con efficacia in tema di sostenibilità. Sul tema della transizione energetica c'è un grave ritardo; non possiamo delegare agli enti locali la programmazione e, soprattutto, la gestione dei singoli progetti. È una visuale che evidentemente non possono avere; è una visione d'insieme che non c'è sui territori. Si corre il rischio di creare dei danni invece di risolverli. Quello che sta accadendo nella mia provincia di Rimini, con l'impianto eolico *offshore*, è molto emblematico È una situazione di grande incertezza.

questo naturalmente genera divisioni e discussioni, sia fra i cittadini che fra le associazioni e, soprattutto, fra gli enti locali coinvolti. È proprio il Pitesai che manca, cioè lo strumento normativo di riferimento per programmare, per mettere i necessari paletti, per valorizzare la sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree del nostro Paese. Paese. Questo strumento avrebbe dovuto dire al privato che, se si punta sulla sostenibilità, allora quel progetto deve essere davvero e che impattare paesaggisticamente, come succede a Rimini, con 50 pale eoliche alte 200 metri a pochi chilometri dalla costa, in una delle spiagge più conosciute e amate del nostro Paese, non è un approccio accettabile sulla via che porta alla decarbonizzazione. che è difficile raggiungere un compromesso fra esigenze contrapposte che puntano sulla sostenibilità, quella della salvaguardia dell'ambiente e quella del paesaggio.

Noi ora dobbiamo assolutamente correre e non possiamo restare fermi su questo obiettivo. Chiudo citando Lucio Anneo Seneca, che dice che non esiste un vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare.

alla quarta votazione il dispositivo da me utilizzato in tribuna non ha rilevato il mio voto favorevole, in quanto il *tablet* si è spento nel momento in cui il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione. Pertanto chiedo che vengano messi a verbale sia la mia presenza che il mio voto.